Signora Presidente, onorevoli senatori, relativamente al divieto di effettuare le operazioni di sfalcio, trinciatura e sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione sino al completamento della fioritura, rappresento quanto segue. Il regolamento UE 2021/2115 prevede che gli Stati membri attivino un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente, alle condizioni ulteriormente specificate nei Piani strategici nazionali della Nelle scelte nazionali del Piano, particolare interesse ha suscitato l'ecoschema 5, «Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori», declinato successivamente nell'articolo 21 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, che disciplina i pagamenti diretti del primo pilastro della PAC. A tal riguardo, rilevo che le superfici sulle quali si praticano le colture di interesse apistico sono superfici a riposo che contribuiscono all'osservanza dell'obbligo del primo requisito delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) della condizionalità rafforzata, corrispondente al 4 per cento delle superfici a seminativi da destinare ad elementi e/o superfici improduttive. Con l'adesione volontaria all'ecoschema 5, sulle predette superfici a riposo è consentito praticare un miscuglio di colture a perdere, il cui mancato raccolto è compensato dal pagamento per l'ecoschema. Per beneficiare delle relative misure nelle superficie a seminativo, l'agricoltore, oltre a possedere titoli su tutta la superficie oggetto di impegno, deve rispettare tre specifici impegni: 1) il mantenimento nell'anno della domanda della copertura dedicata con impianti di interesse apistico spontanea o seminata; 2) il non utilizzo di diserbanti chimici o altri prodotti fitosanitari; 3) la non esecuzione delle operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura, compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. I medesimi impegni, fatta eccezione per il primo, si applicano anche alle coltivazioni di specie di interesse apistico sui terreni investiti con colture arboree, corrispondenti all'altra tipologia di intervento remunerata dall'ecoschema 5. Ciò premesso, riguardo alla richiesta formulata dall'interrogante circa la possibilità di introdurre strumenti derogatori alla durata prevista dal terzo impegno, rilevo che il periodo di interdizione di sfalcio si basa sulla considerazione che i pronubi trovano rifugio ed alimento anche nelle parti secche delle piante e non solo dal solo dal bottinamento dei fiori. Infatti, oltre che dimorare negli steli, alcuni impollinatori svolgono parte del loro ciclo vitale nel terreno. L'obiettivo, quindi, è stato quello di creare delle aree specifiche dove gli impollinatori abbiano la possibilità di svolgere parte del loro ciclo vitale con il minor disturbo possibile. Peraltro, l'ecoschema 5 è un intervento trasversale e generale che trova attuazione in tutto il Paese, a prescindere da differenze di tipo geografico e climatico. Una differenziazione per territorio dei periodi di divieto di sfalcio implicherebbe quindi una notevole difficoltà nel verificare la conclusione del ciclo vegetativo del miscuglio miscuglio delle essenze botaniche e pertanto non è praticabile. Occorre comunque tener presente che, trattandosi di misure volontarie, non è configurabile un regime di deroga, salvo che non intervengano casi e circostanze eccezionali, conclamate e pubblicamente riconosciute, come ad esempio fitopatie a livello epidemico. Riguardo al temuto rischio di incendio rappresentato dall'interrogante, ricordo che i provvedimenti antincendio, attuati solitamente a mezzo di ordinanze locali da parte dei soggetti preposti, sono operanti e applicati a prescindere dagli ecoschemi o dagli interventi di gestione volontari. Mi preme evidenziare, infine, che la durata del periodo e il divieto di eseguire le operazioni in questione sono finalizzati a potenziare la sinergia virtuosa tra gli insetti impollinatori e le piante, alla base del buon funzionamento degli ecoschemi.

devono avere degli aiuti nel portare avanti la loro economia e il loro reddito, con qualcosa che non crei problemi ai loro territori.

La sopravvivenza dell'agricoltura sta proprio nella politica di chi ci governa e di chi riesce a rispondere al grido d'allarme. Questo è stato uno fra i tanti sollevati nelle manifestazioni degli agricoltori e io me ne faccio portavoce. Non si

Signor Presidente, ringrazio gli interroganti per avermi fornito l'occasione per fare il punto sulla situazione degli Istituti penali per i minorenni (IPM) di Treviso e Rovigo, oggetto di massima attenzione da parte di quest'Amministrazione, sin da quando si verificarono i noti eventi del 12 e 13 aprile 2022, che tuttavia andavano correttamente collocati all'interno di un particolare momento storico e ricondotti a problematiche non colte o non adeguatamente trattate nell'ambito dei servizi sociosanitari territoriali, le cui conseguenze hanno poi finito per ricadere sulla giustizia minorile. Il Ministero della giustizia, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), ha da tempo intrapreso uno sforzo considerevole ai fini di garantire la funzionalità e l'efficienza dei propri istituti penali e servizi minorili, nonché di potenziarne l'apparato educativo e socioassistenziale, sia mediante consistenti politiche assunzionali, per far fronte all'atavica carenza di personale, sia mediante lo sblocco degli interventi di edilizia penitenziaria. Il personale civile attualmente in servizio presso gli istituti penali per i minorenni è infatti pari a 254 unità, a fronte delle 343 previste. Tuttavia, a breve si prevede di immettere nel sistema nuove risorse. Entro il corrente mese di ottobre saranno convocati, per la scelta della sede della relativa presa di servizio prevista per il prossimo mese di novembre, i vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 413 unità, da inquadrare nel profilo dei funzionari di servizio sociale; entro il primo trimestre del 2025 si procederà ad assumere ulteriori 91 funzionari della professionalità del servizio sociale. Inoltre, sono state avviate le procedure finalizzate all'assunzione, sempre nel primo trimestre del 2025, di candidati risultati idonei in concorsi banditi da altri enti, mediante lo scorrimento delle relative graduatorie tutt'ora in vigore, con particolare riferimento al profilo amministrativo-contabile e al profilo della professionalità pedagogica. Quanto al contingente del personale di polizia penitenziaria, quello previsto in organico ed assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ammonta complessivamente a 1.613 unità, di cui ne risultano effettivamente in servizio 1.473. Grazie all'entrata in servizio dei neodiplomati del 183° corso di formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria, nel mese di luglio 2024 sono state assegnate al citato dipartimento 133 unità appartenenti al suddetto ruolo, ripartite tra gli istituti penali minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), al fine di potenziare i rispettivi nuclei attualmente presenti sul territorio nazionale. In particolare, presso l'istituto penale per i minorenni di Treviso, ove l'organico del personale del Corpo di polizia penitenziaria previsto era di 35 unità, attualmente risultano presenti 36 unità. unità. La pianta organica è quindi completa. Si consideri inoltre che, in occasione della complessiva riformulazione delle piante organiche di tutti gli istituti e servizi minorili, verrà valutata anche la possibilità di ampliamento della dotazione destinata all'IPM di Treviso. Massimo impegno è stato profuso anche per la parte edilizia della struttura detentiva, che è stata oggetto di manutenzione ordinaria, in attesa che si rendesse fruibile l'IPM di Rovigo. Nell'anno 2023 si è infatti provveduto ad effettuare lavori di ripristino, cogliendo altresì l'occasione per migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle camere detentive e dei servizi annessi. Stanno proseguendo, altresì, i massicci interventi di ristrutturazione e riqualificazione avviati nell'aprile del 2021, necessari ad adeguare il complesso demaniale di Rovigo alle nuove esigenze di questo dipartimento, sotto la direzione del competente provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di stazione appaltante appaltante dei lavori. In particolare, nella seduta del Comitato misto paritetico giustizia/MIT del 31 luglio 2024, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha ottenuto l'assegnazione del finanziamento di 3 milioni di euro per l'esecuzione delle opere in variante programmate. Da ultimo, oltre alle attività finalizzate al potenziamento concreto del personale civile di Polizia penitenziaria finora attuate, il dipartimento si è fortemente e strategicamente impegnato al fine di dare vita a cinque nuove comunità sociosanitarie ad alta intensità terapeutica, dislocate nelle tre macroaree del Nord, del Sud e del Centro e Isole, e di consentirne l'apertura in tempi rapidissimi. Una volta a regime, siffatte strutture concorreranno in modo significativo sia ad alleggerire le circostanziali condizioni di sovraffollamento di alcuni istituti penali minorili, sia a svolgere una funzione deflattiva all'interno delle strutture detentive, riducendo via via quella componente di utenti, prevalentemente i minori stranieri non accompagnati, riversatisi nel circuito penale minorile a seguito delle fattispecie di reato commesse sul nostro territorio. Trattasi di ragazzi provenienti in prevalenza dei Paesi del Nordafrica, spesso poliassuntori di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci, con gravi problematiche comportamentali e che, giunti in Italia, vengono assorbiti da un meccanismo di fisiologica marginalità sociale, aggravata dall'assunzione di sostanze psicotrope, che li conduce alla commissione di reati legati talvolta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non solo, con conseguente assoggettamento a misure penali. Questi giovani finiscono dunque per essere immessi nel circuito carcerario minorile in assenza dei riferimenti familiari e di alternative esperibili, quali comunità educative ad alta intensità sociosanitaria, carenza cronica cui il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sta facendo fronte in accordo con le Regioni, in ragione delle rispettive competenze. non può sottacersi come l'incremento esponenziale dell'utenza minorile degli istituti penali minorili, l'ingravescenza delle devianze giovanili e la gravissima pregnanza lesiva dei fenomeni criminosi che sempre più spesso si verificano abbiano dato causa e, anzi, abbiano richiesto un intervento normativo quale quello attuato giusto un anno fa con l'emanazione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto-legge Caivano, che è intervenuto opportunamente a rafforzare gli strumenti in dotazione alla magistratura minorile, peraltro sostanziati anche da una visione sociale di ampio respiro e da misure a carattere speciale preventivo. Il Ministero della giustizia è ben consapevole e fortemente impegnato sul fronte della riflessione politico-sociale in merito alle cause delle croniche criticità del sistema detentivo minorile, prima fra tutte la risalente mancanza di un'effettiva integrazione sociale di complesse categorie di giovani vulnerabili, fra cui i già menzionati minori stranieri non accompagnati. La strategia prospettica che si è prefissato il Ministero, attraverso le sue competenti articolazioni, comprende un insieme variegato di interventi a vari livelli concettuali ed organizzativi, affinché accoglienza, integrazione e risocializzazione

Signora Presidente, signor Vice Ministro, prendo atto della sua risposta e di quella

Nell'esercizio delle mie prerogative di parlamentare della Repubblica, mi sono recato più volte a visitare l'istituto penale minorile di Treviso, dove ho potuto constatare personalmente le diverse criticità che ho riportato nelle varie interrogazioni parlamentari: sovraffollamento, carenza di spazi adeguati, insufficiente personale della Polizia penitenziaria, mancanza di educatori. questioni cruciali, che solo recentemente hanno iniziato a ricevere qualche timido segnale positivo. Tuttavia, vorrei sottolineare un altro fatto, altrettanto chiaro. Il decreto-legge per scelta del Governo, ha incrementato il ricorso alla detenzione minorile. I dati dell'associazione Antigone parlano chiaro: non solo c'è un dimezzamento dei fondi a disposizione della formazione e del lavoro, ma c'è stato un aumento della detenzione dei ragazzi tra i sedici e i diciassette anni. La vostra politica si riassume in una scelta precisa: aumentare le pene detentive mettere più ragazzi in carcere, ma deve essere chiaro che con la sola repressione, senza investimenti in infrastrutture sociali e scolastiche, non si va da nessuna parte. Ho potuto verificare in prima persona l'impegno e la professionalità degli operatori, ma, nonostante il loro encomiabile lavoro, le carenze strutturali rimangono evidenti, come ho visto anche nel corso dell'ultima visita. La mia prima visita era avvenuta dopo la rivolta che c'era stata

I lavori non hanno fatto altro che ripristinare la situazione preesistente, senza risolvere i problemi. Oggi, allora, voglio essere ancora più preciso in quest'Aula, perché è giusto Grazie

e giovani adulti, a fronte di uno spazio per 12 persone, e questo sovraffollamento comporta la convivenza forzata tra minori e maggiorenni, spesso coinvolti in reati molto diversi. Gli spazi delle celle sono ridottissimi, con bagni di appena un metro quadrato. Lo spazio del refettorio è talmente angusto e limitato che i pasti devono essere serviti in due turni diversi per il pranzo e per la cena. Non esiste uno spazio adeguato alle attività sportive. C'era un campo da calcio, quello della attigua casa circondariale per adulti, che non è più utilizzato da aprile di quest'anno, perché ritenuto A tutto questo si aggiunge la cronica mancanza di personale civile sia in segreteria sia in ragioneria; è vero, sono stati recentemente immessi nuovi agenti di Polizia penitenziaria e cinque nuovi educatori, ho potuto verificarlo, ma non possiamo nasconderci, forti di questi numeri, che la situazione ancora rimane gravemente critica. Per quanto riguarda poi la nuova struttura di Rovigo a cui lei, Vice Ministro, ha fatto riferimento, davvero mi auguro che le promesse si concretizzino, perché quell'istituto potrebbe alleggerire la pressione su Treviso. Tuttavia, chiediamo al Governo di rispettare gli impegni presi e di dotare questa nuova struttura del personale necessario, rendendola operativa il prima possibile. Diversamente, continueremo a trovarci in una situazione di emergenza che non consente il rispetto del dettato costituzionale circa la funzione rieducativa della pena. Signor Vice Signor Vice Ministro, lei è perfettamente consapevole che i nostri istituti penitenziari sono troppo spesso assimilabili a veri e propri gironi danteschi

e al reinserimento sociale dei condannati e deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani. Per queste ragioni, continueremo a vigilare e a incalzare il Governo affinché agisca con decisione e continueremo a farlo nel rispetto delle nostre funzioni parlamentari e nel pieno rispetto anche della nostra Costituzione.

anticipo un comunicato del nostro Dicastero che ristabilisce i giusti equilibri fra i dati comunicati da Antigone e quelle che in realtà sono state le scelte del Ministero sugli investimenti

per quanto riguarda il tema carceri, segnalo che l'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva quesiti in ordine ai molteplici aspetti di criticità che attanagliano il sistema penitenziario e in particolare la carenza degli organici, il tasso di affollamento detentivo e le sue ripercussioni, nonché la manutenzione delle strutture, dando poi specifico rilievo ad alcuni istituti di pena del Paese, quali quelli del distretto umbro. Il tema del sistema carcerario è stato affrontato in molteplici occasioni di risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo, con uno sguardo alla problematica a livello nazionale anche recentemente e sul piano dei singoli distretti e istituti penitenziari, a dimostrazione del fatto che si tratta di questioni cronicizzate e che, nel contempo, questo Governo sta dimostrando di riconoscere, nei fatti, assoluta priorità al sistema carcerario nel suo complesso. Prima di analizzare nello specifico dati e soluzioni riguardanti il distretto penitenziario umbro, è doveroso ricordare che, a livello nazionale, si stanno concretamente impiegando risorse e risposte straordinarie all'emergenza del sovraffollamento, dei problemi strutturali delle carceri e dell'incremento del personale addetto, con soluzioni mirate e lungimiranti che tengano conto di decenni di criticità del settore. Ricordo ancora una volta che il Governo, attraverso il recente decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto carcere sicuro, ricorrendo a una sinergia tra istituzioni, ha lavorato su specifiche direttrici di intervento che mirano ad arginare il sovraffollamento carcerario, a favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione detenzione con la limitazione della carcerazione preventiva e a favorire il trasferimento di categorie più sensibili di detenuti, come i minori e i tossicodipendenti in comunità, potenziando le strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, favorendo così anche l'idoneità di un trattamento differenziato. Tra le disposizioni normative del suddetto decreto-legge, il programma edilizio risulta al centro dell'attenzione, con l'ampliamento della capacità ricettiva delle strutture carcerarie e l'adeguamento agli *standard*. Il complesso intervento sarà curato attraverso la nomina di un commissario straordinario con il compito di attuare in tempi rapidissimi il Piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di Polizia penitenziaria, senza dimenticare le misure per l'incremento del personale del Corpo di polizia penitenziaria attraverso 1.000 assunzioni extra che si aggiungono ad altre 1.000 già disposte lo scorso anno. Ciò che risulta di facile percezione, dunque, è che l'intervento normativo in oggetto, a differenza delle svariate riforme emergenziali che il legislatore ha tentato negli ultimi anni, ha un carattere organico, destinato a incidere profondamente sulla realtà penitenziaria. Gli innumerevoli progetti di edilizia penitenziaria, elencati si muovono inoltre sia sulla direttrice dell'edificazione di nuovi padiglioni e spazi trattamentali e quindi di nuovi posti detentivi, sia su quella dell'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 di strutture penitenziarie già esistenti. Basti pensare che nel Piano di edilizia penitenziaria avviato dall'amministrazione rientra anche la realizzazione di otto nuovi padiglioni detentivi in aree libere e disponibili *intra moenia* presso complessi penitenziari già attivi, il cui finanziamento per 84 milioni è stato inserito negli interventi complementari al PNRR. Come accennato, oltre all'aspetto del miglioramento delle condizioni detentive, ci si è concentrati sullo specifico obiettivo di dare massimo impulso all'implementazione di spazi per attività trattamentali, anche mediante l'ottimizzazione degli spazi detentivi già a disposizione, tanto che nel corso dell'anno 2023 risultano avviati e conclusi interventi per oltre 5.000 metri quadri, tra i quali grande rilievo ha la realizzazione di tre immobili destinati ad attività trattamentali da circa 450 metri quadri cadauno, a completamento dei padiglioni di Lecce, Taranto e Trani. Un'approfondita analisi è stata effettuata attraverso il anche sui numeri della popolazione detentiva; dalle ultime rilevazioni del 7 ottobre 2024 presso gli istituti di pena del Paese sono presenti 61.914 detenuti, di cui 1.341 in regime di semilibertà, rispetto a una previsione regolamentare di complessivi 50.911 posti. Con le citate percentuali di presenza, allo stato attuale non si ravvisano casi di allocazione di detenuti in sofferenza ovvero al di sotto dei limiti di spazio previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e ciò anche perché il monitoraggio nazionale delle presenze è costante. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al 10 maggio 2024 e al 1° ottobre 2024, ha provveduto a effettuare 30 provvedimenti di movimentazione di detenuti che hanno interessato 489 internati e coinvolto le Regioni maggiormente affollate (Lombardia, Lazio, Puglia e Campania), nonché le aree metropolitane di Milano, Napoli e Roma. Nello stesso arco temporale, si è provveduto a disporre lo sfollamento anche delle sezioni di alta sicurezza 3 annesse agli istituti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Prato, Palmi, Augusta, Roma, Rebibbia femminile e Messina femminile. Altro aspetto specifico evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo riguarda il confronto sul numero di volte in cui viene applicato l'isolamento disciplinare in un istituto piuttosto che in un altro, sempre con particolare riferimento al distretto penitenziario dell'Umbria.

Orbene, l'*iter* disciplinare, così come normato, rende particolarmente difficile e sostanzialmente ininfluente il dato statistico sull'applicazione dell'isolamento disciplinare come termine di paragone tra i vari istituti penitenziari. Ancora, si fa riferimento al dato drammatico riguardante gli "eventi critici", riferiti sia agli istituti della Regione Umbria, sia a tutti gli istituti della penisola. Si registra che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2024, negli istituti umbri si siano verificati tre eventi suicidari nel 2022, cinque nel 2023 e uno nell'anno in corso. Drammatici sono anche gli episodi di aggressione agli agenti del Corpo penitenziario e tra detenuti; si registrano 27 episodi nel 2022, 59 nel 2023 55 nel 2024, mentre tra la popolazione detenuta si rilevano 86 episodi nel 2022, 125 nel 2023 e 85 nell'anno in corso. A livello nazionale, si registrano 84 episodi di suicidio nell'anno 2022, 66 nel 2023 e 68 nell'anno in corso. Di fronte alla drammaticità di questi episodi, il Governo si è impegnato concretamente anche su questo versante, potenziando la rete di assistenza psicologica, con progetti di monitoraggio in corso da tempo, e accelerando l'opera di reclutamento di personale adeguatamente specializzato per rispondere alle crescenti esigenze riscontrate tra la popolazione carceraria. Per la prima volta è stata integralmente coperta la pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici (circa 1.100 unità) e il Ministero è intervenuto per il 2024 con risorse a bilancio per i servizi di assistenza psicologica pari a circa 14 milioni di euro, quasi il triplo dell'anno scorso. Altro aspetto cruciale del sistema carcerario è sicuramente quello relativo alle coperture di organico del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, l'atto di sindacato si occupa degli istituti del distretto della Regione Umbria, in cui si rilevano percentuali di scopertura non lontane dal dato nazionale.

La casa di reclusione di Spoleto, a fronte di un organico di 296 unità, conta su una forza presente di 249 unità, inferiore a quella prevista di 47 unità, mentre la casa circondariale di Terni, a fronte di un organico di 262 unità, conta su 201 presenze, con una scopertura dunque di 61 unità. Analizzando nello specifico i recenti incrementi di personale assicurati dal Ministero, si evidenzia che per il ruolo dei funzionari di Polizia penitenziaria, a seguito del concorso del 3 maggio 2024, sia per l'istituto di Spoleto sia per quello di Terni sono state conferite le funzioni di comandante di reparto a due primi dirigenti. A livello nazionale, inoltre, sono stati indetti concorsi il 6 settembre 2023 e il 16 febbraio 2024, rispettivamente per i ruoli di vicecommissario, con 60 posti a concorso, e di sovrintendente, per 293 nuove unità di personale. All'esito delle relative procedure, l'amministrazione terrà conto delle carenze di ruolo specifiche sofferte dagli istituti della Regione Umbria, assegnando un idoneo numero di unità. In ordine alla carenza di agenti/assistenti, l'organico degli istituti penitenziari in questione è stato già incrementato

Entrando nello specifico dei dati forniti dal DAP per ciascun istituto, emerge che presso il carcere di Orvieto risulta coperto l'incarico di direttore, alla stregua dell'area funzionari giuridico-pedagogici, soddisfatta con le cinque unità previste in organico. I funzionari contabili sono presenti in numero di due, a fronte di un organico di tre unità. Con riferimento all'istituto di Perugia Capanne, è stato coperto il ruolo di uno dei due direttori, per la durata di tre anni, mentre è stata avviata la procedura di interpello per l'unico posto vacante. Risulta invece pienamente soddisfatta la pianta organica dei funzionari pedagogici, mentre per i funzionari contabili si registra una sola scopertura su quattro unità previste. Spoleto per l'area dirigenziale risulta coperto nel ruolo del direttore, mentre per i due posti di vicedirettore si è avviata la procedura di interpello il 31 luglio 2024. Quanto ai funzionari pedagogici, l'organico è pienamente soddisfatto con le otto unità previste, mentre i funzionari contabili scontano una sola scopertura. di Terni, su due posti dirigenziali, è dotato del ruolo di direttore per quattro anni ed è scoperto per l'unico posto di vicedirettore. L'area funzionari pedagogici è pienamente soddisfatta, con le sette unità presenti, e per la figura dei funzionari contabili sono Come ribadito in altre occasioni, infine, in tema di organici va evidenziato che il Ministero favorisce da sempre il *turnover* del personale, con una politica di implementazione costante attraverso nuovi bandi di concorso e ampliamento delle previsioni organiche nazionali,

alla situazione davvero invivibile del sovraffollamento - lo sapete - ma anche alla mancanza di organici della Polizia penitenziaria, è un problema di oggi,

Detto questo, in generale, compresa la situazione delle carceri umbre, troviamo una drammatica sottovalutazione.

non lo tenete in considerazione; anzi, praticate una politica carceraria che è l'esatto contrario, in Italia e in Umbria. Diversamente, non si spiegherebbe il fatto che siano aumentati a dismisura i detenuti che dovrebbero stare fuori adesso e non fra un anno o che dovrebbero stare in comunità, se magari sono ragazzi

la civiltà del sistema carcerario di un Paese è allineata al suo sistema di civiltà democratica. Infine,

Donatella Tesei - che probabilmente deve essere un'omonima della candidata alle prossime elezioni come Presidente di Regione - ha annunciato trionfalmente il ripristino del provveditorato regionale, dopo che negli anni i provveditorati erano stati accorpati.

a un mese dalle elezioni arriva l'annuncio della candidata presidente Tesei, della quale non si ricordano in questi cinque anni interventi sulla situazione carceraria.

le vostre responsabilità, di usare il tema delle carceri nella campagna elettorale: i detenuti e il dibattito pubblico non se lo meritano

Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dalle senatrici Fregolent e La Marca, in quanto vertenti sull'analoga problematica della tempistica del rilascio dei passaporti che - com'è noto è da connettere all'incremento delle richieste del documento di espatrio, prodottosi per una pluralità di cause, alcune contingenti, come la fine delle restrizioni post-Covid, e altre di carattere strutturale, come la Brexit. Per far fronte a tale situazione, è stato posto in essere dalle questure uno straordinario impegno organizzativo, articolato, tra l'altro, in interventi di potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione degli uffici e nella ristrutturazione del sistema di prenotazione *online*. In particolare, tale sistema di prenotazione è stato implementato con una sezione cosiddetta agenda prioritaria per la gestione delle urgenze per coloro che hanno necessità di partire nei successivi trenta giorni, per motivi di studio, lavoro, salute o turismo, consentendo al cittadino di prenotare un appuntamento presso l'ufficio passaporti in tempo utile all'effettuazione del viaggio. Il nuovo sistema prevede inoltre, in caso d'incapienza dell'agenda prioritaria, la possibilità di presentazione immediata della richiesta agli sportelli della questura, senza che occorra un appuntamento. Le misure adottate hanno consentito di raggiungere risultati molto positivi. Infatti, dall'inizio dell'anno in corso sono stati emessi più di 2,347 milioni con un *trend* in aumento rispetto al 2023, quando, nei primi nove mesi dell'anno, ne erano stati emessi circa 2,07 milioni. In relazione In relazione alle specifiche situazioni segnalate negli atti di sindacato ispettivo, rilevo che a Parma l'organico dell'ufficio passaporti è stato incrementato ed è attualmente di dieci operatori. Le misure intraprese, come accennato, consentono attualmente l'effettuazione di prenotazioni caratterizzate da urgenza mediante il ricorso

con il titolo che viene reso disponibile nei tempi richiesti dall'utente. Nella Provincia di Parma, nel corso del 2024 e fino al 2 ottobre, sono stati consegnati complessivamente circa 22.000 passaporti. Anche nella Provincia di Cagliari, tra le misure organizzative adottate dalla questura, vi è il potenziamento dell'ufficio passaporti, che è passato dall'iniziale organico di cinque operatori, previsto nel 2022, a quello attuale composto da quattordici dei quali assegnati in via permanente e quattro aggregati a rotazione, provenienti da vari uffici della Polizia. L'incremento del personale ha consentito non solo di ampliare i servizi di sportello per l'acquisizione delle istanze, ma anche la programmazione di aperture straordinarie di due pomeriggi della settimana, con con modalità *open day*, rendendo possibile ricevere e definire complessivamente circa 600 pratiche a settimana. Dal mese di marzo scorso è stata inoltre raddoppiata la disponibilità degli appuntamenti prenotabili in calendario e, contestualmente, si sono ridotti i tempi di consegna del documento. Sempre dal mese di marzo è stata attivata la procedura dell'agenda prioritaria con la disponibilità sul Comune di Cagliari di 10 *slot* al giorno e dal successivo mese di aprile ulteriori 10 *slot* giornalieri sono stati previsti anche in ambito provinciale. In tutta la Provincia, alla data del 30 settembre scorso, sono stati stampati complessivamente circa 28.000 passaporti. Su un piano più generale, un ulteriore e decisivo contributo per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini è rappresentato dal progetto Polis, che consente di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente agli sportelli delle Poste italiane senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il Governo, dal marzo scorso, ha dato avvio al progetto e lo sta progressivamente estendendo su tutto il territorio nazionale, con l'attuale coinvolgimento di 213 sportelli dislocati in altrettanti Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Dal mese di luglio è consentita anche l'accettazione delle istanze di rilascio di passaporto a favore dei minorenni, per i quali non sussistono provvedimenti giudiziari che dispongano in ordine alla responsabilità genitoriale o tutoria. Aggiungo che lo scorso mese di giugno è stata siglata un'ulteriore convenzione tra il Ministero dell'interno e Poste Italiane che consente di estendere la modalità di presentazione delle istanze presso gli uffici postali anche nei centri urbani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il servizio, che allo stato coinvolge sperimentalmente le città di Roma, Bologna, Cagliari e Verona, sarà progressivamente esteso all'intero territorio nazionale. nelle prime tre sedi pilota (Bologna, Verona e Cagliari) sono state presentate circa 3.530 istanze di rilascio passaporto presso gli uffici postali, di cui 2.102 definite con l'emissione del titolo. Le iniziative illustrate vanno quindi nell'auspicata direzione della semplificazione procedurale e dell'efficientamento complessivo del sistema. In tal senso, si sono registrati apprezzamenti sia da parte dei cittadini sia dell'organizzazione del comparto turistico. Da ultimo, si assicura che l'amministrazione continuerà a monitorare la situazione affinché il servizio di rilascio dei passaporti avvenga con la massima celerità su tutto il territorio nazionale.

in cui si mettevano a disposizione 70 passaporti; 240 persone in fila d'attesa, i numeri esauriti già nel primo giorno - il *click day* era di due giorni consecutivi - e cittadini che

un incremento, in un certo senso sono positivi. Mi chiedo, però, cosa occorra ancora per rendere tutto molto più veloce, dato che la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un *trend*.

sforzarsi per far migliorare la pubblica amministrazione in questo settore, posto che dubito che da qua

scarso funzionamento della qualità della relazione tra il Parlamento e il Governo. Ho apprezzato la sua risposta: ci ha dato atto che ci si sta muovendo e, molto onestamente, ripetuto più volte l'avverbio "progressivamente". Ecco, vorremmo che questo "progressivamente" diventasse subito o immediatamente o si desse

economiche legate a questo mondo. Nel biennio 2022-2023 i *tour operator* e le agenzie hanno denunciato 300 milioni di mancati introiti, pari a 167.000 viaggi annullati perché i clienti non sono riusciti ad avere il passaporto in tempo. Com'è stato correttamente ricordato, parliamo anche di enormi difficoltà nell'ottenimento della carta d'identità elettronica che, benché in minima parte, aiuterebbe o concorrerebbe a risolvere il problema. Questi dati sono stati forniti da Confindustria e Assoviaggi, ma sono molti Confindustria e Assoviaggi, ma sono molti i *tour operator* che hanno continuato a lamentare la situazione. Le sei città che sono state monitorate un anno dopo la presentazione di quest'interrogazione, sempre «Il Sole 24 Ore», confermano l'odissea della prenotazione anche sulle piattaforme *online* nei capoluoghi di Regione: tre mesi a Roma e a Milano, mentre in in sei città non ci sono disponibilità, salvo il canale delle urgenze, nonostante un aumento dei rilasci avvenuto nel 2023, di cui lei ha riferito e di cui le si dà atto. Tuttavia, ottenere il passaporto in Italia è davvero una missione impossibile,

la necessità di risolvere tutto questo. Lei ha anche citato l'efficacia di Polis, il progetto sperimentale. Da quanto risulta, ci sono situazioni in cui funziona abbastanza bene e altre, invece, in cui le cose ancora non funzionano, ma i cittadini sono tutti uguali e devono avere tutti lo stesso diritto, quello di muoversi e viaggiare. È un diritto che va ugualmente garantito a tutti, quindi occorre fare di più. Occorre fare in modo che il Paese dia risposte all'altezza dei tempi. Chi mi ha preceduto ha ricordato la necessità di investimenti importanti, soprattutto nell'informatizzazione e nello snellimento della burocrazia. Fare un passaporto non può essere un'odissea. Devono

riconoscendo che è un diritto umano fondamentale. Lo scopo di questa Giornata è quello di accrescere la consapevolezza dei problemi di salute mentale in tutto il mondo, vuole anche ricordare che bisogna rendere più concreta e accessibile ogni attività a sostegno della salute mentale, cominciando dal contrasto a ogni tipo di discriminazione e dalla lotta dalla lotta contro lo stigma che ancora accompagna le persone che, in qualche modo o in qualche momento della propria vita, soffrono di una condizione di disagio psichico o di malessere psicologico. Nel corso del 2023 le persone con problemi di salute mentale che sono state prese in carico

- il disagio mentale è molto più diffuso: sono almeno due milioni i cittadini italiani che non hanno avuto alcun accesso alle cure e sono proprio i dipartimenti di salute mentale, che in questi anni sono andati via via

con 150 incontri in tutta Italia. Grazie al sostegno di cittadini, volontari e operatori sanitari e amministratori,

Il fine è diffondere un segnale forte e visibile di vicinanza e condivisione prima di tutto alle persone che soffrono di problemi mentali o di disagio psichico o psicologico e poi ai loro familiari, che spesso pagano il prezzo da soli, in solitudine, facendosi carico,

di problemi di salute mentale. Si tratta anche di un segnale di vicinanza alle tante meritevoli associazioni impegnate a promuovere la cultura della salute mentale. Vorrei concludere il mio intervento ricordando che questo 10 ottobre è straordinariamente importante e significativo per il nostro Paese e per l'Europa, perché proprio quest'anno ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia. Franco Basaglia. Egli ha rivoluzionato il mondo della salute mentale e ha restituito dignità alle persone che soffrivano di problemi psichici, fino al fino al momento in cui finalmente si aprirono le porte di quei manicomi in cui venivano confinati, dimenticati, discriminati e abbandonati. Proprio per essere all'altezza della straordinaria rivoluzione che Franco Basaglia ha determinato con la sua intuizione e il suo lavoro, credo che oggi vi sia la necessità di dare risposte molto più importanti e di ritornare a investire, immaginando non di tornare all'apertura dei manicomi, ma di creare

accolte, aiutate e sostenute nel pieno rispetto della loro dignità e del benessere loro e dei loro familiari. ringrazio, senatrice Zampa, anche per averci ricordato che l'eredità di Franco Basaglia è ancora un tema in pieno svolgimento e da svolgere.

delle due arterie principali che lo costeggiano, la SS 249 e la SS 45-*bis*, che ultimamente sono state interessate sempre più frequentemente da importanti e seri eventi franosi, che stanno mettendo in allarme tutto il nostro territorio, minando altresì la sicurezza e l'incolumità di chi transita attraverso quelle strade. Ricordo che il lago di Garda è uno dei motori turistici più importanti in Italia, cuore d'Europa per il turismo, e che, a fronte delle tre interrogazioni - questa è la quarta - che ho sottoposto a lei, Ministro, e al Ministero che lei guida, ad oggi non ho ancora ricevuto risposta. Nel corso degli approfondimenti che abbiamo fatto, è emerso che le barriere paramassi sono obsolete, nei tratti della Gardesana, e non riescono più a intercettare i massi che cadono sulla strada. Molte risalgono agli anni Sessanta e agli anni Settanta. Quindi sono qui a interrogarla in merito. Parallelamente a questa tematica abbiamo la questione della ciclovia del Garda, dove ci si è impuntati a voler creare un anello che passa attraverso dei tratti molto importanti, pericolosi e inaccessibili. Qualche settimana fa è iniziata la traforazione della prima galleria Cantone dal lato Veneto, proprio per permettere ai ciclisti di attraversare la galleria - si tratta di uno dei tratti più pericolosi, una delle strade più pericolose d'Italia - ben sapendo che alla fine la ciclovia si arresterà e i ciclisti si riverseranno sulla Gardesana, creando ancora più pericolo a chi transita su quella statale. Sapendo che il decreto del 2018 considera la possibilità di utilizzare trasporti alternativi alla pista ciclabile, quali i battelli sostenibili, sono qui a chiedere: quali interventi strutturali urgenti sono stati pianificati o già eseguiti in seguito alle frane occorse; se sono stati previsti fondi straordinari per l'adeguamento delle barriere paramassi e la manutenzione delle infrastrutture esistenti; quali azioni di coordinamento il Ministero intenda intraprendere con le autorità locali e regionali alla luce della mancata progettazione avanzata della ciclovia del Garda; la sospensione della traforazione e l'utilizzo di strumenti di trasporto alternativi. PRESIDENTE. Il ministro

dalla collega, e ovviamente di dare rassicurazioni ai cittadini sull'attenzione che il Governo e tutti gli enti territoriali coinvolti dedicano gli aspetti legati alla sicurezza. Il progetto della ciclovia - non entro nel merito delle strade, risalenti agli anni Sessanta, e rispondo di quello che stiamo facendo oggi con questo Ministero e questo Governo Governo - risale a un decreto interministeriale del gennaio 2022. Esso è stato il frutto di un lungo confronto tra i Ministeri al tempo interessati e tutti gli enti territoriali, aperto anche alla partecipazione di associazioni ambientaliste di cicloturisti.

di Toscolano Maderno, Limone sul Garda e Salò, per un investimento complessivo di 480.000 euro, con la posa di barriere paramassi conformi agli *standard* europei. Sulla SS 249, la Provincia autonoma di Trento ha stanziato, nel corso degli ultimi anni, mediamente oltre 100.000 euro all'anno per le opere di mitigazione del rischio di crolli rocciosi. Nell'ultimo triennio sono stati realizzati tre interventi di somma urgenza per ripristinare l'agibilità e mitigare il rischio di crolli nel tratto compreso tra Torbole e il confine con la Provincia di Verona, per un investimento complessivo di circa 500.000 euro. Per quanto attiene alla situazione delle barriere difensive sulla Gardesana orientale, relativamente alla sponda occidentale, la Provincia autonoma di Trento ha sviluppato un progetto pari a 7 milioni di euro, che individua gli interventi per la messa in sicurezza del versante soprastante la ciclovia. Tale progetto è esecutivo e in fase di approvazione e a breve verrà messo a gara. Relativamente invece alla sponda orientale, si procederà analogamente. Per quanto attiene al tratto veneto da lei citato, la società Veneto strade ha confermato di aver svolto tutti gli approfondimenti necessari alla verifica delle condizioni, anche in riferimento agli interventi nella galleria Cantone, nei Comuni di Torri del Benaco e Malcesine, due tratti soggetti a fenomeni erosivi. Sono previsti interventi di consolidamento del fronte attraverso la posa in opera di reti protettive e barriere paramassi. Con tutte queste misure, il tracciato della ciclovia assicurerà adeguate garanzie in termini di sicurezza dai crolli di versante, con la creazione di un percorso dedicato ai pedoni e ai ciclisti lungo le due arterie. Il valore aggiunto di questa ciclopedonale è quello di un anello ciclabile della lunghezza complessiva di circa 166 chilometri, nell'assoluto e ovvio rispetto degli *standard* di sicurezza per i lavoratori e i futuri utenti.

dalla sua risposta, che anzi, ritengo una vera presa in giro nei confronti del territorio che sono chiamata a rappresentare. Le ricordo che lei è il Ministro dei trasporti e che è suo dovere garantire la sicurezza e l'incolumità di tutte le persone che attraversano le nostre strade, e quindi non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I ciclisti hanno diritto di attraversare in sicurezza le nostre strade e il nostro territorio tanto quanto gli automobilisti non vogliono investire le persone. Sappiamo benissimo che quella nel territorio tra Navene e Torbole, che ha citato, è una delle strade più pericolose d'Italia e che, costruendo quel tratto nella galleria Cantone, la ciclovia si interromperà e si riverseranno sulla Gardesana ancora più ciclisti di quelli che abbiamo attualmente. Richiamo quindi la sua responsabilità e il suo dovere di Ministro dei trasporti e non dei disastri, perché noi non vogliamo morti per ulteriori frane. Non vogliamo morti per ciclisti investiti. E chiediamo di rivalutare la sospensione della ciclovia, che costerà un patrimonio al nostro territorio. Abbiamo il dovere di tutelare la reputazione che abbiamo a livello internazionale con il lago di Garda. State distruggendo spiagge che sono il motivo per cui i turisti vengono da noi. Quindi, chiedo al Ministro di contattare i responsabili locali e regionali, che poi fanno anche parte del suo partito. **Saluto Saluto la delegazione dell'Università di Teramo, guidata dal Rettore, che oggi in Senato inaugura il *master* di

il decreto-legge che ripartisce il Fondo complementare al PNRR sono stati stanziati alla Regione Campania più di 500 milioni di euro. Con il decreto interministeriale del 28 febbraio 2023 dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia sono stati stanziati fondi per oltre 103 milioni di euro per opere immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali della Campania. Con il decreto del maggio 2024 il Ministero delle infrastrutture ha stanziato più di 84 milioni di euro per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario della Campania; tali risorse erano destinate a sette nuovi treni. La parte di rete ferroviaria Campania di proprietà della Regione è affidata in gestione all'Ente autonomo Volturno, e in particolare alle ferrovie isolate Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, e altre tratte campane, in un territorio che interessa milioni di utenti locali e migliaia di turisti che raggiungono i luoghi di cultura e della tradizione campana. I fondi citati comprendono anche risorse per rimodernare la ferrovia Circumvesuviana e il tratto ferroviario della valle di Suessola, che riscontrano evidenti carenze infrastrutturali e gestionali. Negli ultimi anni si è avuta una progressiva riduzione del numero delle corse giornaliere, del numero dei treni e delle corse disponibili, per i quali risulta carente anche la manutenzione e che sono insufficienti ad accontentare le esigenze di un'intera utenza, sempre più insoddisfatta, in un territorio dove le ferrovie rappresentano una fondamentale integrazione agli altri sistemi di mobilità del territorio. Signor Ministro, le chiediamo quale sia lo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dal Ministero delle infrastrutture per il complesso sistema delle ferrovie della Campania. le chiediamo, signor Ministro, se abbia individuato le responsabilità sulle carenze nel servizio e nella rete infrastrutturale, e come intenda intervenire per porre le basi per migliorare lo stato delle ferrovie campane e il servizio a favore dei pendolari, degli utenti e dei turisti.

Sul piano infrastrutturale sono finanziati, a valere sul Fondo complementare PNRR - come lei ricordava - cinque interventi gestiti dall'Ente autonomo Volturno, dipendente dalla Regione Campania per il potenziamento delle ferrovie regionali, per un investimento complessivo di 546 milioni di euro. Rispetto a tali interventi sono state già aggiudicate le procedure di gara e sono in corso di esecuzione i relativi contratti. In particolare, per l'adeguamento agli *standard* di sicurezza delle gallerie, il potenziamento della tratta Castellammare-Sorrento e la digitalizzazione degli impianti della circolazione dei mezzi, la conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026. La fornitura dei treni per il trasporto pubblico locale dovrebbe invece completarsi entro giugno 2025.

e la Benevento-Bosco Redole. L'avanzamento complessivo dei lavori delle due opere procede regolarmente, secondo programma, nel rispetto dei termini del PNRR. Questi investimenti si inseriscono in un più ampio quadro di finanziamenti per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza della rete ferroviaria regionale campana. Ne cito alcuni, non tutti, per non rubarvi troppo tempo: con il PNRR sono stati destinati alla Regione Campania 287 milioni di euro, alcuni dei quali per l'acquisto di 10 treni elettrici a zero emissioni, 84 milioni per la fornitura di altri sette sul nuovo capitolo REPowerEU e i restanti 109 milioni sono destinati al potenziamento e ammodernamento della linea Cancello-Benevento. Per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, la Regione Campania è assegnataria di 145 milioni di euro. Completo il quadro con i fondi per lo sviluppo e la coesione, per i quali Ente autonomo Volturno si è visto assegnare altri 240 milioni di euro per il miglioramento dell'accessibilità alla stazione di Afragola per il nodo di Napoli-Piazza Garibaldi e per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'intero sistema del trasporto pubblico locale campano. Se poi questi soldi si tramuteranno in fatti e miglioramento del servizio, ovviamente sarà competenza del Ministero che ho l'onore di guidare garantire un attento monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, perché nemmeno un euro dei cittadini campani assegnato a Regione Campania vada sprecato nella realizzazione di queste importanti opere. *(Applausi)*.

predisposto e indirizzato al Governo. I motivi sono evidenti, ma ritengo comunque opportuno ripercorrere in maniera anche molto sintetica gli eventi dell'ultimo periodo, partendo dai mesi estivi, in cui abbiamo registrato una condizione allarmante del settore ferroviario proprio nel suo periodo cruciale, ovvero quando al normale flusso si va ad aggiungere quello straordinario legato al turismo. Siamo al 9 luglio, stazione di Centola, un incidente ha compromesso per giorni il traffico sulla dorsale tirrenica con limitazioni, ritardi e cancellazioni; due giorni dopo, 11 luglio, altro incidente di un treno merci, questa volta a Parma, ha causato feriti e sospensione della circolazione; 18 luglio, sulla linea Trieste-Venezia, un vagone si stacca dal treno merci perdendo lungo la linea quanto stava trasportando, ovvero autovetture, e causando ritardi e cancellazioni. Sempre il 18 giugno, un grave incidente tecnico a un treno Freccia, questa volta nei pressi di Ancona, provoca cancellazioni e ritardi oltre le cinque ore. Il giorno successivo, siamo al 19 luglio, il caos questa volta è a Firenze, a Rovezzano, dove un danno all'alimentazione della rete elettrica mette in crisi per l'intera giornata tutto il sistema di Alta velocità nazionale

errori umani e sistemi che non funzionano e restituiscono quotidianamente un sistema trasportistico al collasso. Ciò di certo non aiuta la sua scelta, signor Ministro, di mettere mano al codice degli appalti, introducendo il cosiddetto subappalto a cascata, che va a svilire il requisito Signor Ministro, le chiedo se lei non ritenga opportuno avviare quanto prima un piano straordinario di manutenzione ordinaria delle ferrovie, esattamente come sembrerebbe le sia stato suggerito dall'Autorità di

l'interrogazione presentata, che mi permette di ringraziare le migliaia di lavoratrici e lavoratori di Ferrovie dello Stato, RFI e Trenitalia che anche in questo momento, mentre stiamo parlando in Senato, stanno lavorando su oltre 1.100 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana per garantire sicurezza; investimenti e cantieri che, purtroppo, devono andare a recuperare anni e anni di mancata manutenzione e mancati investimenti precedenti.

portandoli da 2,2 a 2,8 miliardi di euro nel recente aggiornamento. La manutenzione ordinaria è svolta prevalentemente da personale di RFI al fine di mantenere in piena efficienza gli impianti e le apparecchiature. Nel quadriennio 2020-2023 sono stati eseguiti 60 milioni di ore di manutenzione ordinaria, pari al 65 per cento del monte ore totale di manutenzione. Riguardo agli investimenti di manutenzione straordinaria, segnalo che nel primo semestre del corrente anno 2024 è già stato effettuato il rinnovo di ben 550 chilometri di binari, 480 deviatoi e terminati 50 interventi manutentivi su ponti e gallerie. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria si aggiunge quella eccezionale necessaria nei casi in cui eventi imprevedibili, alcuni dei quali da lei ricordati, rendano indispensabili interventi al fine di garantire la sicurezza nell'esercizio ferroviario. In risposta alle richieste di chiarimenti al Ministero sulle ragioni dei disservizi, il gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato, con riguardo all'evento dello scorso 2 ottobre, che l'evento si è manifestato dopo il danneggiamento di un cavo da parte di un'impresa appaltatrice (quindi non subappaltatrice). Il danneggiamento ha comportato la disalimentazione della cabina di media e bassa tensione. Sono quindi entrati in funzione i sistemi di *backup*, che solitamente garantiscono la continuità del servizio, ma che, per cause che RFI sta accertando - e se qualcuno ha sbagliato, rovinando la giornata di lavoro a migliaia di persone, ne pagherà le conseguenze - nel caso di specie hanno portato all'attivazione delle misure di protezione elettrica. Sull'accaduto, come detto, RFI ha nominato una commissione d'indagine con l'obiettivo di accertare cause e responsabilità dell'evento. A seguito delle evidenze rassegnate dalla commissione, sono in corso di attuazione i conseguenti provvedimenti gestionali e organizzativi. Concludo ringraziando nuovamente le migliaia di lavoratori, operai, tecnici e ingegneri che ogni giorno garantiscono la mobilità a centinaia di migliaia di cittadini italiani in questo straordinario Paese.

manutenzione non effettuata negli ultimi anni - ricordando però che nel contratto di programma che annualmente viene aggiornato da RFI e Ministero vengono stanziati soldi per la manutenzione. Io non posso assolutamente ritenermi soddisfatta da una risposta del genere, così come dal suo operato. Mi dispiace dal suo operato. Mi dispiace dirlo ma, per ironica analogia con il sistema dei trasporti che dovrebbe garantire, lei arriva in quest'Aula estremamente in ritardo, sciorinando tra l'altro una serie dei suoi soliti elenchi. Le rispondo, con dati alla mano,

di questi ha raggiunto dei ritardi superiori alle due ore. Signor Ministro, nel periodo 2023-2024 abbiamo registrato 5.000 ore di interruzioni ferroviarie e più di 6 milioni di euro di richieste di rimborsi di biglietti in più,

come l'idea del subappalto, che comunque resta un problema del codice degli appalti. Signor Ministro, mi viene da chiederle se lei si ritiene soddisfatto di come sta facendo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; se le risulta sufficiente il tempo che dedica al suo lavoro nel Ministero, pari a tre o quattro ore al mese; in ultimo, se ci fosse un altro soggetto al suo posto, Ministro, di fronte alla disastrosa

fino a trenta minuti. Se consideriamo le condizioni meteo, lei si renderà conto di qual era la situazione di tutti gli utenti che oggi usavano il treno nella mia Regione.

deve concordare che questo sistema non può reggere. Non possiamo avere un sistema ferroviario colabrodo, che ogni giorno porta i cittadini italiani a non sapere se e quando partirà il treno. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) segnala oltre 10.000 interruzioni della linea all'anno,

anni. Noi le chiediamo non solo le motivazioni di questi guasti, ma anche un piano straordinario. Le chiediamo di venire in quest'Aula un giorno intero a raccontare tutto quello che avviene su tutte le reti italiane, a raccontare e ad ascoltare.

è controllare le acque che il buon Dio ci manda in terra. E, quindi, almeno il controllo della pioggia non dipende dalla nostra volontà. Dipende dalla nostra volontà, invece, vigilare sulle società concessionarie come Rete

il loro lavoro. A beneficio collettivo, faccio alcuni esempi sperando di non annoiarvi perché prima ho dato dei dati su numeri, finanziamenti, tratte ferroviarie, tempi di esecuzione, ma mi si è detto di non fare le liste. D'altronde, se un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non dettaglia investimenti, periodi e fine lavori, non fa il suo mestiere. Siccome voi ricordate anche una presunta mancanza di trasparenza sugli investimenti ferroviari per il PNRR, ne ricordo alcuni che riguardano i pendolari che l'Alta velocità: corridoi TNT, potenziamento dell'Alta velocità e miglioramento delle reti regionali usate dai pendolari quotidianamente. Tra le principali grandi opere in corso da Nord a Sud con i cantieri aperti oggi, ricordo la nuova linea Napoli-Bari; il raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania e della tratta Catania-Fiumetorto sulla Catania-Palermo; il passante di Firenze, opera straordinaria ultimata la quale non ci sarà più interruzione sull'Alta velocità nel caso di un guasto sulla linea, anche di un treno merci; il quadruplicamento della Brescia-Verona-Vicenza e della Fortezza-Ponte Gardena; il Terzo Valico dei Giovi e la nuova linea di Alta velocità Battipaglia-Romagnano. Altri interventi riguardano i raddoppi delle tratte ferroviarie Fabriano-Albacina, Ripalta-Lesina, Lunghezza-Guidonia, Campoleone-Aprilia, Codogno-Cremona-Mantova e Decimomannu-Villamassargia. Ricordo che nei piani di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria finanziata con fondi PNRR sono stati stanziati non uno, ma 22 miliardi di euro di investimenti, di cui il 40 per cento focalizzato al Sud. A questi vanno aggiunti ulteriori interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti regionali

con riferimento agli investimenti sulla flotta regionale che usano studenti e pendolari tutti i giorni, ci sono 6 miliardi di euro investiti per l'acquisto di 1.061 treni di nuova generazione, consentendo una diminuzione netta dell'età media dei convogli che abbiamo ereditato, soprattutto al Sud. Quindi, come ultima riflessione, le misure compensative per gli utenti richiamate dall'interrogante per i disagi dello scorso 2 ottobre fino ad oggi sono state lavorate ed evase con esito positivo 4.788 richieste di indennizzi e rimborsi in base a quanto previsto dalla normativa. Ne approfitto per ringraziare per l'ennesima volta lavoratrici e lavoratori che garantiscono un eccellente servizio ferroviario a migliaia di utenti sulle ferrovie italiane ogni giorno, con 1.100 cantieri aperti e si tratta di un *unicum* a livello continentale.

Non sono invece per niente soddisfatto della circostanza che lei non risponde a una domanda molto semplice: quando nasce la responsabilità di un Ministro?

il 45 per cento dei voli, con oltre un milione di richieste di risarcimento del danno. Allora, signor Ministro, qui il tema è la sua responsabilità: lei che cosa intende fare oltre a chiedere informazioni? Qui c'è una proprietà transitiva delle informazioni: noi le chiediamo a lei, lei le chiede a RFI e RFI le chiederà alla società subappaltatrice. Allora cancelliamoli i Ministeri, facciamo soltanto società per azioni e vediamo cosa si fa. Lei ha una precisa responsabilità. Risponda a questo Parlamento al più presto. Venga qui a spiegare perché il sistema dei trasporti è andato in tilt. So che lei ha molti impegni perché è anche vice presidente e segretario del suo partito. Ma, se vuole continuare a fare il Ministro, risponda di ciò di cui lei è responsabile; altrimenti quel chiodo, quando glielo portano, lo può utilizzare per appenderci le scarpe.

ma si configura come elemento essenziale per garantire che tutti i cittadini possano esercitare in completa sicurezza il "diritto alla mobilità", previsto dall'articolo 16 della Costituzione; il crollo del "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, ha provocato 43 vittime e molti feriti, con centinaia di famiglie che hanno subito un enorme danno per l'incuria di un'opera infrastrutturale in esercizio nonostante il suo elevato stato di decadimento, per evidenti responsabilità dei soggetti che dovevano gestire l'opera, ma anche per una mancata attenzione da parte del sistema nazionale rispetto alla gestione di un sistema autostradale dato in concessione; fornire un sostegno alle vittime di incuria infrastrutturale costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria, anche in virtù della diffusa percezione che determinati eventi, sebbene colpiscano direttamente solo alcuni cittadini, a ben vedere offendono l'intera comunità civile; sarebbe, dunque, ragionevole prevedere che eventi dannosi collegati a cedimenti totali o parziali di infrastrutture di rilievo nazionale, conseguenti a forme di incuria derivanti da errori o inadempienze in sede di progettazione e manutenzione, possano, quali che siano le responsabilità accertate e i risarcimenti previsti in sede giudiziale, configurare un intervento da parte dello Stato, anche in virtù del fatto che spesso i tempi dei processi penali sono irragionevolmente lunghi e le spese giudiziarie ingenti, si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine sostenere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, le vittime di eventi dannosi derivanti dell'incuria nella gestione e manutenzione della rete infrastrutturale. il quesito affronta un tema di grande rilievo etico e sociale non solo per la Liguria, ma per l'intero Paese. La tragedia del Ponte Morandi, che ha scosso l'Italia intera, ci impone di agire in una duplice direzione, sulla quale abbiamo impegnato i nostri mesi in questo Governo; da un lato, la vicinanza non solo morale dello Stato italiano ai familiari di chi ha perso la vita in quel tragico incidente; dall'altro lato, l'impegno a intensificare i controlli, che evidentemente in passato sono mancati, gli interventi di manutenzione straordinaria e i grandi investimenti per rafforzare la sicurezza della nostra rete infrastrutturale, autostradale e stradale. Con questa consapevolezza, da ultimo, nei mesi di luglio e agosto scorso, abbiamo lavorato insieme al Ministero dell'economia e delle finanze per trovare una soluzione al tema del riconoscimento di forme di sostegno concreto alle vittime e ai familiari del crollo del Ponte Morandi. Lo abbiamo fatto in raccordo intenso con il Comitato «Ricordo vittime del Ponte Morandi», che ringrazio, e insieme con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che avevano presentato disegni di legge sul tema. Il testo risultante da questo lavoro è stato affidato alla Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, che proprio ieri ha chiuso l'esame del provvedimento con la votazione degli emendamenti della relatrice e l'approvazione degli articoli. Il provvedimento istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2025, più 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il fondo sarà destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale. Per ogni vittima è prevista una donazione *una tantum* e l'attivazione di specifiche misure, incluse quelle integrative di sostegno al reddito per le famiglie in condizioni di bisogno. Inoltre, come avviene per i figli delle vittime del terrorismo, prevediamo la possibilità di accedere alle assunzioni dirette da parte dello Stato e la concessione di borse di studio annuali riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi. Ci tengo a sottolineare lo spirito di questo provvedimento, che ha visto lavorare tutti i Gruppi politici presenti in quest'Aula (e li ringrazio). Tutti siamo consapevoli che non esiste cifra al mondo che possa ripagare chi ha perso i propri cari, ma è giusto e doveroso che lo Stato risponda con norme di civiltà sociale e giuridica per ricordare e sedimentare nella memoria del nostro Paese un principio fondamentale: nessuno può e deve morire per l'incuria derivante da errori di progettazione o per la mancata manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali. *(Applausi)*.

si intende il riuscire a rialzarsi dopo un fatto grave più forti di prima. Oggi, grazie allo sforzo di tutti - come lei ha appunto ricordato - per arrivare ad un testo condiviso, senza distinzione di maggioranza, di opposizione, di schieramento politico politico o altro, il modello Genova ha preso una nuova forma che ci vede tutti uniti nel dare risposte concrete. Ritengo che questo sia il miglior esempio che le istituzioni possono dare nell'affrontare, come in questo caso, una tragedia. investimenti sul piano infrastrutturale. La Regione Liguria ricopre un ruolo strategico nello scenario logistico europeo; le opere infrastrutturali sul territorio incrementeranno crescita e competitività e sicuramente non dovranno più essere causa di incidenti e tragedie. Tutte le opere in corso di realizzazione sono una straordinaria leva di sviluppo e offrono una grande occasione di riscatto per la Regione e per tutto il Paese. Grazie alla sua azione ministeriale e al Governo stiamo sbloccando infrastrutture attese da decenni e continueremo a farlo, contro l'immobilismo e a beneficio di tutti i liguri e dell'Italia intera. Grazie, Ministro.

lei ha preso il posto del suo predecessore, che ha avuto qualche vicissitudine personale. Siccome a noi non interessa quello che fa un Ministro nella camera da letto, ma interessa molto quello che fa un Ministro quando si riveste e va in ufficio, dobbiamo prendere atto del fatto che Sangiuliano, il suo predecessore, ha scelto per la guida di Ales, la principale azienda di servizi culturali di questo Paese, con tantissimi lavoratori assunti e con tantissimi appalti, una persona il cui *curriculum* è impresentabile e ridicolo. Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale (quella che ci vende sul *curriculum* è robetta) e ha come grande pregio, agli occhi di chi lo ha nominato, quello di essere stato assessore ai servizi sociali in quota Fratelli d'Italia a Frosinone, che è un ruolo importantissimo, ma non propriamente connaturato e collegato ad Ales. Egli ha poi spiegato in tutte le trasmissioni televisive che si forma guardando i video di Giorgia Meloni, che è una cosa anche interessante. Non so a quale video di Giorgia Meloni egli faccia riferimento. Forse, che so, al video sulle accise in cui Giorgia Meloni dice "elimineremo le accise" (poi non lo ha fatto) o al video in cui Giorgia Meloni dice "noi sulle trivelle non accetteremo mai (…)!" (forse quello) o forse al video in cui Giorgia Meloni diceva di voler uscire dall'euro. In ogni caso, non risulta al sottoscritto un *tutorial* di Giorgia Meloni, che sarebbe sicuramente efficace, su come si governa una società chiamata Ales. Allora la domanda è: questa presidenza è stata scelta in nome di una valutazione di merito o in nome dell'amichettismo, come io penso? Siccome lei sta facendo un *repulisti* (leggo) di quelli di prima, le domando se per caso intenda fare *repulisti* anche sul buon Tagliaferri. Cito: «Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia delineante questo - «alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale» il risultato è duplice e speculare. Sono le sue frasi di ieri in Commissione. Io trovo interessante sia la citazione, non contenuta qui, di Hegel; sia quella, che trovo, di Luciano Floridi; sia una citazione, che ho visto solo io, di Monicelli, Tognazzi e del conte Mascetti, a proposito della sua strategia culturale. Signor Ministro, le domando: che ci azzecca con Hegel e la rivoluzione permanente dell'infosfera globale un NCC di Frosinone alla guida di un'azienda dei servizi culturali? Almeno lei mi risponda a voce, come sa fare lei, e non come ha fatto il "chiodo Salvini" qualche minuto fa.

prometto da oggi che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi.

cultura*. Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto, che mi offre l'occasione per illustrare e chiarire, mi auguro definitivamente ma a questo punto senza illusioni, i tratti salienti della vicenda in oggetto. Anzitutto è opportuno ribadire questo: Ales - Arte, Lavoro e Servizi SpA è una società *in house* a partecipazione pubblica totalitaria che svolge prevalentemente attività funzionali alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Essendo una società a controllo pubblico, Ales è soggetta alla disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) - che immagino il senatore Renzi conoscerà bene - e, per quanto ivi non espressamente derogato, alle norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. Il suddetto testo unico, in particolare, con riferimento all'assunzione e alla questione del personale delle società a controllo pubblico, rimette alle società stesse la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Nello specifico, per rispondere a uno dei quesiti posti, Ales, durante l'attuale presidenza, ha sempre seguito per il reclutamento del proprio personale procedure di valutazione comparativa, imparziali e trasparenti, in conformità alla legge e ai principi sopra richiamati, senza avallare dunque modalità non rispondenti ai requisiti del merito e della competenza. Da quanto risulta a questo Ministero, peraltro, anche le assunzioni fatte dalla struttura e dagli uffici preposti durante i mesi della presidenza Tagliaferri non hanno suscitato reclami o impugnative di qualsivoglia genere da parte di alcun partecipante alle procedure di individuazione e reclutamento, svoltesi secondo modalità chiaramente disciplinate e prestabilite, né rilievi sono pervenuti a tal proposito dagli organi di gestione e di controllo della società medesima, che non sono a Frosinone (che pure mi sembra cubi circa

ascoltate bene, se potete - di non voler autorizzare il sospetto che tale insistito e allusivo rumore di fondo intorno a lui sia dovuto alla mal riposta illusione che Tagliaferri medesimo venga distratto dal compito affidatogli

Da parte nostra si conferma qui non soltanto la regolarità formale della procedura di designazione, ma altresì il valore professionale del dottor Tagliaferri, il quale, oltre ad aver ricoperto diversi incarichi, vanta una indiscussa e duratura esperienza manageriale.

per evitare che continuasse lo spreco di fondi pubblici che causava, altrimenti questa sarebbe stata una buona piattaforma da dove trasmettere un racconto poco avvincente. Chiudo, senza l'ombra di alcun *arrière-pensée*, cogliendo l'occasione per riconfermare la mia stima professionale nutrita nei confronti di Antonella Manzione, già capo dei Vigili urbani di Firenze, scelta nel 2015 alla guida dell'Ufficio affari legislativi della Presidenza del Consiglio dall'attuale interrogante e allora *premier* Matteo Renzi, che a suo tempo mi lusingai di difendere in pubblico dall'inaccettabile accusa di aver trasformato Palazzo Chigi in un comitato d'affari paesano. *(Applausi)*.

Signor Presidente, non ho ancora iniziato la risposta. Immagino che possa iniziare adesso il tempo. PRESIDENTE. Faccia la sua replica. RENZI *(IV-C-RE)*. Se lei non mi interrompe e lo dice ai suoi colleghi di partito, le sono grato. abbiamo visto tremare non tanto semplicemente la sua mano, ma la sua voce. Al di là delle battute sulle capacità cognitive, senz'altro limitate del sottoscritto, ma in grado di far conseguire al medesimo una laurea in tempi decenti, cosa che auguriamo possa accadere anche a lei, il punto centrale è che lei non ha risposto alle domande su Ales. Però a questo punto, guardi, Presidente, togliamo il vino dai fiaschi. A me del *gossip* non interessa niente, a me interessa sapere chi è stato assunto e come, chi ha preso i soldi e come. Sono i soldi del pubblico. "Con la cultura non si mangia" non vuol dire che qualcuno può mangiare a parte, quindi se voi entro una settimana ci rispondete bene, altrimenti procediamo nelle sedi istituzionali altre. Il punto politico, visto che ho ancora un minuto, è che sì, sicuramente, è stata "prematurata con scappellamento a destra come fosse antani" la risposta monicelliana del Ministro, ma il punto chiave è che lei non ha dato una risposta di politica culturale. Voi avete messo uno che non ha un *curriculum* adatto per stare lì e lo avete difeso e avete messo in campo una polemica contro una consigliera di Stato, la dottoressa Manzione, che non soltanto aveva tutti i titoli per stare lì e che trovo offensivo che lei citi, ma che addirittura ha svolto un servizio - sì, al Paese - in quegli anni in cui lei ci difendeva. Le segnalo che facevo il sindaco di Firenze, non di Lignano, che è importante almeno quanto la sua Frosinone per la gestione dei beni culturali; in quella fase lì lei, caro lei, caro ministro Giuli, anziché venire qui e dialogare con noi, è venuto a farci la lezioncina, che noi, da uno che dava del patriota a Vladimir Vladimirovich Putin, non prendiamo. Vi misureremo sull'attività dei Beni culturali. Vi chiediamo la risposta alle domande entro una settimana e vi invitiamo a scoprire la gentilezza e l'umiltà nel posizionarsi non di fronte all'interrogante, ma di fronte al Parlamento della Repubblica, che *pro tempore* la ospita come Ministro.

- Premesso che: la cultura è l'anima di una nazione, sancisce le identità nazionali e ne incarna i valori e i principi fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la democrazia e il pluralismo; dal 19 al 21 settembre si è tenuta, al palazzo Reale di Napoli, la riunione dei ministri del G7 Cultura, presieduta dall'Italia, nel corso della quale è stato ribadito il ruolo centrale della cultura per le nazioni, per i popoli e per le comunità, come bene e responsabilità dell'umanità, strumento facilitatore del dialogo interculturale e intergenerazionale, come generatore di attività come generatore di attività economica e di posti di lavoro; i Ministri ivi riuniti hanno affermato, per la prima volta a livello internazionale, la necessità di rispondere tempestivamente agli interrogativi, non solo di natura etica, posti dall'intelligenza artificiale ed esaminare il suo impatto sul ruolo degli artisti, dei creativi, degli operatori tutti della cultura; in merito, nella dichiarazione ministeriale "La cultura, bene comune dell'umanità, responsabilità comune", sottoscritta al termine dei lavori, si afferma la volontà di perseguire in campo culturale "una trasformazione digitale inclusiva, incentrata sull'uomo, che sostenga la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, massimizzi i benefici e gestisca i rischi, Pertanto, chiedo alla sua cortesia quali siano stati gli intendimenti del Ministero che ha l'onore e l'onere di guidare in relazione alle conclusioni del G7 che ha presieduto, in particolare con riferimento agli effetti e all'impatto dell'intelligenza artificiale nel campo culturale; di quali proposte si fa portatrice l'Italia e quali sono gli obiettivi che il Governo intende perseguire per garantire la centralità dell'uomo e della sua creatività.

di esporre alcuni degli esiti conclusivi dei lavori del G7 cultura di Napoli, al quale non ha partecipato la Russia, evidentemente impegnata a godersi un miliardo di accordi commerciali siglati nel 2016 da un Governo allora rappresentato

Renzi, non ho colto esattamente le parole, ma colgo invece il modo non corretto di replicare da parte sua. Prego, Tra le altre questioni, abbiamo affrontato nodi cruciali, come il sostegno all'Africa per la valorizzazione delle sue risorse culturali, nello spirito del Piano Mattei, o la tutela dell'identità culturale dell'Ucraina e del suo patrimonio. Una parte significativa dei lavori è stata dedicata all'intelligenza artificiale che il Governo italiano, su indicazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha individuato tra i temi chiave della Presidenza italiana del G7. I Ministri della cultura del G7 hanno concordato di perseguire nei settori culturali e creativi una trasformazione digitale inclusiva e incentrata sull'uomo, che favorisca la crescita economica e lo sviluppo sociale sostenibile, nel rispetto dei diritti umani e dei valori democratici. L'intelligenza artificiale sta infatti aprendo nuove strade per la conoscenza (basti pensare alla decifrazione in corso dei papiri di Ercolano), ma comporta anche dei rischi rischi sul piano etico (quando i processi creativi sono sottratti al controllo umano e i contenuti generati sono utilizzati per disinformare o creare campagne d'odio) e sul piano economico e sociale (quando, ad esempio, le opere della creatività umana, da un romanzo a un brano musicale, vengono utilizzate senza riconoscere agli artisti il diritto d'autore). La dichiarazione di Napoli è il primo documento G7, uno dei primi a livello internazionale, che affronta vari profili dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla cultura e sulla creatività. Parte da un assunto semplice: la creatività è un'abilità posseduta solo dagli esseri umani. Come dice Federico Faggin, lo scienziato italiano che ha inventato il primo microprocessore, solo l'intelligenza umana ha coscienza. A Napoli c'è stato accordo sul fatto che le società che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare le legislazioni vigenti in materia di proprietà intellettuale, prendere adeguate precauzioni per tutelare i diritti dei creativi e garantire qualità e trasparenza dei dati utilizzati per allenare le macchine. In merito vi segnalo che, su iniziativa italiana, i Ministri della cultura del G7 si sono impegnati a promuovere l'identificazione e l'autenticazione dei contenuti culturali interamente o parzialmente generati, modificati o alterati da sistemi di intelligenza artificiale, riprendendo la proposta normativa del Governo italiano recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, attualmente all'esame di quest'Assemblea, che specificamente interviene nel campo del diritto d'autore e dei servizi dei *media* audiovisivi. Con l'Unione europea discuteremo su come utilizzare il potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura, anche per favorire lo sviluppo

e nell'audiovisivo è stata prevista di regola l'esclusione dai costi eleggibili ai fini del *tax credit* produzione delle spese sostenute per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle prestazioni creative e artistiche. I medesimi principi sono stati riportati anche in ulteriori decreti in fase di predisposizione, *in primis* il decreto relativo al credito d'imposta per l'attrazione di investimenti internazionali. Signor Ministro, mi dichiaro completamente soddisfatto dalla sua risposta e sono certo che, per la sua qualità, sarà capace di continuare il lavoro e di realizzare la visione in ambito culturale che questo Governo ha già messo in campo, segnando una netta discontinuità con la storia degli anni pregressi, di una certa intelligenza - lo dico in italiano, perché in latino risulterei l'equivalente dell'onorevole Renzi in inglese e di nomine che sono state cannibalizzate, insieme ai finanziamenti pubblici che queste persone hanno ricevuto, salvo oggi fare un moralismo che, per pulpito, è assolutamente inaccettabile. Non so dove debbano formarsi i nuovi operatori della cultura italiana. Io dico che certamente non devono formarsi sui video di chi aveva promesso di lasciare la politica se avesse perso un *referendum.*

vorrei utilizzare questi minuti di fine seduta per porre alla sua attenzione l'esigenza di richiedere un'immediata calendarizzazione

converrà con me sul fatto che in questa sede e in questo momento noi dobbiamo esprimere tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai militari italiani impegnati nel contingente della Forza di in queste ore è stato oggetto di un attacco da parte dell'esercito israeliano. *(Applausi)*. Riteniamo indispensabile che si mettano in atto subito tutte le iniziative tendenti a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo di questa natura, in considerazione del fatto che l'argomento era stato sollevato nel corso delle audizioni con i ministri Tajani e Crosetto la scorsa settimana nelle Commissioni congiunte esteri e difesa e che il ministro Tajani ci aveva fornito delle garanzie in tal senso. Evidentemente non è accaduto quello che ci si prefigurava potesse accadere. Chiediamo che il Governo intervenga subito e, se è possibile anche che il ministro Tajani si rechi in Libano per sgombrare il campo rispetto a questa

con il Libano, che hanno visto coinvolti i nostri militari. Penso che sia ineludibile, ancora una volta, ricordare l'azione dei nostri soldati, quanto hanno lavorato per salvare la pace in questi anni, il loro impegno ed esprimere quindi tutta la nostra solidarietà rispetto a quello che è accaduto in queste ore. Penso, altresì, che sia stata importante anche l'immediata risposta del Governo. Leggo dalle agenzie che il ministro Crosetto ha chiamato il Ministro israeliano alla difesa non solo per chiedere conto di quello che è accaduto, ma anche per sottolineare che quanto accaduto non solo non può essere ripetibile, ma è oggettivamente inaccettabile: anche e soprattutto quando parliamo con amici,

perché quando accadono queste cose, quando si mette a rischio e a repentaglio chiunque, ma soprattutto i nostri soldati che in questi anni hanno lavorato per la pace, ritengo che non ci sia mai un minuto da perdere e sono contento che il Ministro non l'abbia perso.